ai destinatari le concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica. Infatti, i destinatari delle concessioni non hanno potuto ancora avviare le attività trasmissive a causa della mancata riassegnazione e dell'esercizio delle stesse dalle reti private eccedenti. Tale sentenza ha sancito che l'Italia, nel mancato riassegnamento delle frequenze, ha violato quanto disposto dalla direttiva della della Comunità europea 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. proprio perché la menzionata direttiva 2002/21/CE costituisce la base normativa su cui viene adottata la direttiva 2007/65/CE, della quale si dà delega al Governo per il recepimento con la presente legge comunitaria 2008, e considerato che la direttiva 2002/21/CE viene richiamata dalla direttiva 2007/65/CE al considerando 14, se non si procede ad adeguare le concessioni televisive come disposto dalla Corte,

Rispetto al merito della questione, poi, vorrei chiarire qual è il punto, molto delicato. Parliamo di inserimento di prodotti. Per i colleghi che non seguono la materia è un'espressione un po' ambigua. In realtà, dovremmo dire

all'interno della narrazione del film o della trasmissione in questione. Lo spettatore non si accorge che quella è una pubblicità perché magari c'è l'attore che fuma una determinata sigaretta di cui si inquadra il pacchetto o usa un altro tipo di prodotto. Quindi, si tratta di una pubblicità che sta dentro processi manipolativi... Senatore Fleres, le posso assicurare che il senatore Vimercati sta facendo un intervento interessante sui messaggi occulti nelle trasmissioni televisive. So che lei è particolarmente sensibile al tema.

per applicare questa direttiva. Il Governo italiano di allora, il Governo Prodi, l'aveva interpretata in modo restrittivo; ora vedo che c'è un orientamento diverso. Chiedo pertanto che venga interpretata in modo restrittivo almeno relativamente ai minori, perché i minori esposti alla pubblicità occulta sono particolarmente indifesi. Penso, per esempio, a tutte le questioni relative ai disturbi alimentari: le merendine che vengono proditoriamente inquadrate come *product placement* sono particolarmente dannose per lo sviluppo dei nostri bambini. Così come sono credo da evitare gli inserimenti nei programmi religiosi, sociali, civili. Per questo chiedo alla maggioranza una particolare sensibilità proprio su tale aspetto relativo ai minori e a questa tipologia di programmi.

da parte dei colleghi della maggioranza che, almeno sul tema dei minori e sulle questioni delle trasmissioni religiose e civili, penso saranno d'accordo con noi.

è piuttosto chiara sull'argomento che nel gergo viene chiamato del *product* *placement*, cioè dell'inserimento del marchio di un prodotto durante una narrazione

l'applicazione italiana della direttiva - e purtroppo in materia televisiva non è la prima volta - allarga moltissimo le maglie di tale recepimento e quello che è nella direttiva un caso di eccezione diventa invece un caso di normale amministrazione. Vorrei far presente, colleghe e colleghi, un fatto di attualità. Credo che la bellissima serie televisiva sulla figura di Di Vittorio

di programmi che promuovano la solidarietà e che sconfiggano discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, nazionalità, religione, convinzioni personali, disabilità, età ed orientamento sessuale e che non incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Insomma, non voglio fare un elenco, peraltro testuale e che si rintraccia nel Capo 2-*bis* della direttiva, che per

un po' di buon senso nella normativa italiana, che non tocca temi di cui io stesso mi occupai tanti anni fa, come ad esempio l'affollamento degli *spot*.

di recepimento della direttiva, il quotidiano andamento del nostro sistema mediatico. Chiedo quindi di rispondere su questo emendamento e prego prego di accoglierlo, perché è un emendamento chiarificatore ed indispensabile per quel buon senso della comunicazione

il ministro Ronchi, in Commissione, ha dichiarato, sulla mia riflessione sulla tutela dei minori in TV, di condividere pienamente le dichiarazioni del senatore Di Giovan Paolo sulla tutela dei bambini nei programmi televisivi, tutela che presuppone un giudizio morale e pre-politico.

«Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008, impegna il Governo a considerare l'applicazione della direttiva 2007/65/CE» - quella che si riferisce alla TV senza frontiere - «come il primo passo per una riflessione complessiva sui programmi di informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. In particolar modo studiando gli accorgimenti legislativi che, tenendo conto delle specificità delle piattaforme analogiche, digitali, satellitari e IPTV (via Internet), possano contemperare il diritto a comunicare, l'iniziativa economica» - perché non vogliamo certo deprimere l'iniziativa economica in questo settore - «e imprenditoriale e il prioritario diritto educativo/informativo dei minori, ipotizzando anche una specifica disciplina legislativa di proposta e tutela radiotelevisiva a favore dei minori». Ho ascoltato il dibattito, ho ascoltato la replica del Ministro e abbiamo fatto una proposta che potrebbe essere un passo avanti per tutti. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, accetterei la proposta che viene dalla relatrice di trasformarlo nell'ordine del giorno il cui testo

parere del Governo

2007/64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, si prevede la definizione delle procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento, predisponendo strumenti per la risoluzione delle controversie, sia a livello giudiziale che stragiudiziale. presentato dal Gruppo Italia dei Valori, introducendo la possibilità di agire anche in forma collettiva per la risoluzione di dette controversie, vuole introdurre anche per la materia dei servizi di pagamento la possibilità di intentare azioni collettive risarcitorie, che la finanziaria del 2008 aveva introdotto per la violazione del codice del consumo e a tutela degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

e quindi le ulteriori tutele fossero inserite a monte, nella direttiva, e quindi fossero obbligatoriamente identiche per tutti gli Stati che applicano la normativa. Altrimenti, l'estensione diventa insidiosa perché apparentemente è un'ulteriore tutela, ma di fatto crea una condizione di disparità tra le imprese.

che prescrive appunto l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile. Noi chiediamo solo l'applicazione di una normativa,

Marinaro esprimo parere contrario, perché è proprio contrario allo spirito della direttiva che è quello di diminuire comunque le spese.

Per quello che mi riguarda, direi che i servizi pubblici sono praticamente già esclusi da questa direttiva, per cui forse non sarebbe bene farli rientrare all'interno di questa direttiva. Per quanto quanto riguarda i finanziamenti di compensazione che non possano essere qualificati aiuti di Stato, senatore Di Giovan Paolo, bisogna vedere con quali criteri e in quali modi. Penso sia un criterio difficile da far accettare dall'Unione

definiti nei prossimi mesi, una volta predisposti dal Governo, possano essere trasmessi agli organi parlamentari (in questo caso alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato) per una loro

che vanno nella direzione di esplicitare alcuni principi, senza nulla togliere all'impianto generale di definizione dei criteri a cui dovrà ispirarsi il recepimento della direttiva.

nell'attuazione della direttiva siano garantiti i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati nel nostro Paese. Questo vale per le imprese italiane ma anche, ovviamente, per quelle straniere che vengono da fuori ad operare nel nostro Paese e che non possono, da questo punto di vista,

Analogamente, insisto sull'emendamento 41.203. Noi chiediamo di aggiungere al testo predisposto dalla Commissione e concordato con il Governo un esplicito riferimento alla necessità di elencare le attività di servizi che vi rientrano e non un generico riferimento

aveva già avviato un lavoro di *screening*, di pulitura di tutte le normative preesistenti nel nostro Paese che in qualche modo contrastano con il recepimento della direttiva in e su cui lo stesso tavolo delle Regioni si era espresso positivamente negli scorsi mesi. Dunque, con questo emendamento intendiamo recuperare questo lavoro e contribuire ad una «pulitura» delle norme in contrasto con la

Con l'ultimo emendamento che abbiamo presentato, il 41.207, chiediamo di sopprimere il comma 3 che prevede che questa delega non abbia spese accessorie a carico dello Stato.

è che ci sia un recepimento meramente formale della direttiva. In assenza di risorse adeguate è difficile agire, dato che parliamo di una direttiva che si inquadra nell'ambito della più vasta cornice di rilancio dell'economia comunitaria, che parte dalla strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato dei servizi più competitivo, più unitario, più transnazionale, al fine di incoraggiare una crescita economica uniforme in tutta l'Unione europea. Lo scopo della proposta è quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono la libertà di stabilimento tra le imprese, anche nel settore dei servizi. Da questo punto di vista è importante, ad esempio, la previsione, che noi condividiamo, della realizzazione di alcuni

sanno che questa è una riflessione fatta dall'Associazione europea degli enti locali e regionali, cui appartengono i Sindaci di tutti i colori, i Presidenti di Provincia di tutti i colori e stiamo attendendo, dopo la direttiva

sono disposto ad accettare i cambiamenti proposti dalla relatrice: riguarda lo stesso argomento e naturalmente ho già indicato quali sono i cambiamenti, facendo riferimento alla proprietà da parte degli enti locali come responsabilità politica oggettiva.

Scusi l'interruzione, senatore Di Giovan Paolo. Invito a fare attenzione o a consentire a chi vuole di fare attenzione: ci sono dichiarazioni in cui si accetta di ritirare emendamenti e di presentare ordini del giorno e non si può lavorare in queste condizioni.

di far sì che, oltre a quello dei Ministri interessati, vada acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni rappresentative degli enti locali?

ed invito i colleghi a votare stando al loro posto e con la propria tessera: evitiamo questi spiacevoli episodi, che non hanno alcuna scusante se non la peggiore giustificazione soggettiva.

Prendiamo atto della sua precisazione che, comunque, aveva già espresso dando il parere

è giustificato dal fatto che la decisione in oggetto costituisce uno dei pilastri della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, in quanto tratta di un delicatissimo problema di criminalità organizzata. Nello specifico, visto che è una battaglia che - nostro

la pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace, che corrisponda alle aspettative dei cittadini ed alle esigenze degli Stati membri, e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. L'Italia, adoperandosi a recepire la decisione quadro con decreto legislativo specifico, può contribuire a costituire uno spazio europeo di cooperazione giudiziaria in materia di polizia.

per dare legalità e sicurezza e combattere le mafie, la criminalità organizzata, la 'ndrangheta, la camorra, l'illegalità. Credo, quindi, che anche in Europa la nostra azione di Governo, anche con gli amici dell'opposizione, sia stata quella di condurre un'azione forte contro tutte le criminalità.

ma su un tema così importante come quello della lotta alla criminalità non accetto, personalmente, politicamente e come rappresentante del Governo, qualsiasi tipo di digressione. Questo Governo, questa coalizione, questa maggioranza hanno come priorità la lotta alla criminalità in Italia e in Europa. Lasciamo stare la demagogia e la campagna elettorale in quest'Aula.

e le autorità giudiziarie in materia penale. Il Capo IV è stato approvato all'interno delle Commissioni anche su indicazioni e con emendamenti del Partito Democratico e dell'opposizione ed era volto a favorire la lotta contro la criminalità sotto tutti i punti di vista. All'interno del Capo IV e dell'articolo 46 si fa riferimento in particolare allo scambio di informazioni ed attività addirittura con le *intelligence*, con le forze di polizia; si interviene in materia di sequestri, di riconoscimento delle sentenze penali. L'emendamento 46.100 riguarda una precisa decisione quadro del Consiglio del 2008 che concerne in maniera specifica la criminalità organizzata.

ad una decisione quadro che concerne la criminalità organizzata contraddice la politica stessa annunciata, ma soltanto sulla stampa ed in televisione, dal Governo. Invitiamo questo Governo e questa maggioranza a condurre una lotta contro la criminalità concretamente in sede parlamentare. Il Partito Democratico voterà quindi sicuramente a favore

Le confische afferenti le attività di criminalità organizzata di stampo mafioso sono regolate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

di determinare la responsabilità da reato degli enti anche i delitti contro l'industria e il commercio. Con questa modifica sarebbe possibile confiscare non soltanto il bene mobile e immobile, ma anche il profitto derivante dal diritto.

Senatore Pedica, accetta l'invito al ritiro

favorisce il reinserimento dello stesso nell'ambito sociale. In secondo luogo, la decisione quadro permette anche di poter alleggerire il carico degli istituti detentivi italiani se, da quanto risulta da cifre del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, questi detenuti

a dire che nel caso in cui vi siano detenzioni ingiuste o illegittime siano previsti strumenti giuridici per riparare a questo fatto antigiuridico.

l'Aula del Senato sta approvando con grande e colpevole ritardo una legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2008 e che potrebbe costringere il Governo a ricorrere a provvedimenti urgenti per adeguarsi agli obblighi europei in scadenza. In occasione dell'esame del provvedimento in titolo abbiamo rilevato una preoccupante inclinazione da parte dell'Italia a subire procedimenti di infrazione. Diverse sono le procedure che rischiano di giungere ad una seconda sentenza di condanna con cui la Corte di giustizia impone anche sanzioni pecunarie che comporteranno comporteranno pesanti oneri economici per le casse dello Stato. I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente, della fiscalità, degli appalti e riguardano le carenze a livello regionale e locale. Le nostre proposte si sono concentrate in particolare sul tema della parificazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Abbiamo ritenuto opportuna l'introduzione del principio di flessibilità e di volontarietà per la permanenza nel luogo di lavoro a favore di quelle donne che sono impegnate nella cura dei figli o dei congiunti riconosciuti disabili gravi o dedite alla cura degli anziani. Nell'esercizio della delega affidata al Governo per recepire una direttiva in materia televisiva sta particolarmente a cuore del nostro Gruppo il fatto che venga predisposta un'adeguata protezione dei diritti dei minori nelle trasmissioni televisive. Il ritardo accumulato e la necessità di adempiere agli impellenti

un lavoro che si protraeva da troppi mesi. Si deve comunque riconoscere che, nel lasso di tempo intercorso, maggioranza e opposizione hanno giocato di sponda e che tanti degli articoli contenuti nel testo sono frutto di mediazione, discussione e posizioni condivise. Il lavoro della 14a Commissione è stato proficuo ed ha permesso di approfondire alcune materie importanti, come quella della liberalizzazione dei servizi nel mercato comunitario o, ancora, quella della parità di retribuzione e di trattamento. Come vice presidente della Commissione, vorrei ringraziare la presidente Boldi per la correttezza dimostrata nella gestione della discussione e per l'approccio di apertura ai suggerimenti provenienti dall'opposizione. Vorrei ringraziare poi

ma anche nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo, i cui suggerimenti, espressi tramite la competenza co-legislativa, l'Italia dei Valori ha inteso raccogliere, ad esempio aumento delle garanzie di sicurezza in materia di detenzione delle armi, come consigliato dalla stessa Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

rimpatri, seccamente introdotta nella legge comunitaria con un emendamento del Governo. In proposito, richiamo qui l'impegno del nostro Parlamento al rispetto e all'applicazione delle decisioni europee secondo il principio della sussidiarietà. Vorrei

che si attesta a 164, 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario; proprio su questo punto il lavoro di squadra tra maggioranza e opposizione dovrebbe essere dovrebbe essere più stretto non solo per il buon nome del Paese, ma anche per le sue finanze in quanto, in caso di inottemperanza alle pronunce della Corte, può essere imposto il pagamento di una somma forfetaria e di una penalità di mora. di mora. Ciò anche per sottolineare come la bocciatura del nostro emendamento all'articolo 25, con il quale si chiedeva di recepire integralmente ciò che la Corte di giustizia aveva stabilito in merito alla cosiddetta legge Gasparri e all'assegnazione delle frequenze radiotelevisive, appaia

i cittadini. Cari collegi del centrodestra, noi queste cose le ricorderemo anche durante le campagne elettorali, da qui fino al 2013.

televisiva vince una gara contro un'altra emittente televisiva (Rete 4). Nello stesso tempo, infatti,

di una procedura d'infrazione, come ha ricordato più volte anche in Commissione la presidente Boldi, ma per un rinvio pregiudiziale, ha comunque valenza fondamentale per il nostro ordinamento,

Suggerisco, quindi, alla maggioranza di fare un conto economico prima di rifiutare il contributo che l'Italia dei Valori vi ha dato attraverso emendamenti ed invitandovi ad una riflessione tutti insieme su argomenti che riguardano problemi di ordine nazionale. Lo ripeto: oltre la rete televisiva, la criminalità organizzata e l'ordine pubblico, queste sono materie che vi ricorderemo da qui al 2013.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ringrazio innanzi tutto la relatrice, senatrice Rossana Boldi, per l'accurato lavoro svolto in Commissione e in Aula. Ricordo inoltre quelle che - a nostro avviso - costituiscono le direttive comunitarie di maggior impatto per l'importanza degli argomenti trattati: ad esempio, la direttiva 2006/54 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il provvedimento concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è quello del 15 agosto 2009, con possibilità di proroga di un anno, «ove necessario per tener conto di particolari difficoltà», che mi auguro non si verifichino, per cui la delega possa esercitarsi nei tempi previsti. Di non minore importanza è l'attuazione della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che prevede l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole - previsti dalla direttiva - ad altre tipologie di finanziamento e il rafforzamento dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Testo unico bancario per contrastare le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Con la sentenza del 25 luglio 2008, la Corte di giustizia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 226 del Trattato, ha dichiarato che l'Italia, non avendo provveduto alla corretta trasposizione dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante prescrizioni minime di sicurezza e salute e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima. In particolare, la Commissione europea ha rilevato che la normativa italiana di recepimento ha limitato l'obbligo di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute alle ipotesi di cantieri la cui entità presunta sia superiore a 200 persone al giorno, e di quelli i cui lavori comportano rischi particolari, sebbene l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57 non consentisse alcuna restrizione in merito alla designazione dei coordinatori medesimi. Pertanto, in considerazione della necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, emessa all'esito della procedura d'infrazione comunitaria, n. 205 del 2002, e al fine di precisare la portata della norma, rendendola pienamente conforme al diritto comunitario, è intervenuta la presente legge. Va sottolineata, inoltre, la notevole portata economica dell'articolo 41 che reca una delega al Governo per dare attuazione alla direttiva servizi che avrà un forte impatto sull'ordinamento, in quanto dovrà assicurare la necessaria omogeneità della regolamentazione dei servizi, esclusi quelli di interesse generale come definiti dallo Stato, rispetto ai criteri imposti dalla direttiva, al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori di servizi anche attraverso l'istituzione di sportelli unici nazionali. Tra le modifiche approvate dalla Commissione, rispetto ai criteri di delega proposti dal Governo, è stato introdotto anche il principio finalizzato a garantire l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie ai danni dei cittadini italiani nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri. Il Capo IV riguarda invece le decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Gli articoli da 46 a 49 dettano disposizioni per dare attuazione alle decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e di *intelligence* tra le autorità degli Stati membri, e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Per dare solo qualche dato utile, ricordo che metà delle persone transitate per le nostre carceri nel 2007 era straniera (per una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro), un reato su tre è commesso da clandestini, ma solo uno su nove fra quelli identificati viene realmente espulso. Grazie a questo provvedimento e alle successive norme e accordi internazionali volte a dar seguito ad esso, si potrà far scontare la condanna di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea nel Paese d'origine, anche senza il consenso dell'interessato, attualmente obbligatorio per legge. Questa possibilità viene introdotta con un emendamento del Governo (che anticipa il conferimento della delega per l'attuazione della decisione quadro dell'Unione europea del 2008/909/GAI di tre mesi fa) rafforzato da una raccomandazione volta a garantire l'impegno del Governo in questa direzione, che consentirà l'adozione del decreto legislativo relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, senza dover attendere l'entrata in vigore della comunitaria 2009, che presumibilmente non avverrà prima dell'inizio del prossimo anno. Si tratta di un provvedimento che può costituire un ottimo deterrente per chi viene a delinquere nel nostro Paese, contando su un sistema carcerario decisamente meno duro rispetto a quello dei Paesi di provenienza. Ogni Stato dell'Unione potrà far scontare nello Stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria, così che Paesi ad alto tasso di immigrazione comunitaria, come l'Italia, vedranno alleggerirsi il peso dell'esecuzione delle sentenze emesse, secondo un modello già sperimentato su base bilaterale e prescindendo in varie ipotesi dallo stesso consenso della persona trasferita. Quella di Bruxelles è una decisione quadro che dovrà essere recepita obbligatoriamente da tutti Paesi membri dell'Unione entro il 5 dicembre 2011, ma per quanto ci riguarda la situazione d'emergenza, che si è creata con le bande di delinquenti calate in Italia dai Paesi dell'Est, ha consigliato di accelerare i tempi: presto saremo pronti. Poi bisognerà solo attendere il recepimento della norma da parte degli altri Paesi europei, per rispettare il principio della reciprocità. Nell'interesse comune ci aspettiamo, in particolare dalla Romania, fattiva collaborazione per rendere operativo l'accordo in tempi brevi. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentati del Governo, facendo null'altro che il proprio dovere, questo ramo del Parlamento nella discussione, tardiva e travagliata, sulla legge comunitaria 2008 e sulla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha confermato vistosamente l'insofferenza di questo Governo a stare dentro un quadro di regole condivise. Un Governo che anche quando partecipa ai numerosi vertici europei rimane concentrato sugli ambiti nazionali con chiusure e rigidità di altri tempi e dimostra palese disinteresse verso le strategie che vengono attuate a livello europeo. A questo proposito sono rivelatrici, ministro Ronchi, le sue dichiarazioni sull'Europa dei bollini, oppressiva e burocratica, che sommate al difficile rapporto di questo Governo con le istituzioni politiche europee, a partire dalle misure in materia di sicurezza e immigrazione, a quelle sugli aiuti di Stato, all'affidabilità delle scelte economiche nazionali, alle misure sulla competitività e il mercato interno, alla posizione sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dimostrano un ripiegamento nazionale su una concezione liberal-mercantile dell'Unione europea. Anche rispetto all'informazione istituzionale prodotta dall'Unione europea per le elezioni europee avete preso le distanze per miope provincialismo. Cari colleghi, così facendo si rischia di danneggiare noi stessi e il processo di integrazione europea. Infatti, trascurare il legame tra dimensione comunitaria ed interna rischia di rivelarsi una tragica colpa per l'interesse nazionale, in particolare nell'attuale fase di crisi. Per contare e pesare nel mondo ed in Europa bisogna farsi promotori non di sole misure italiane, ma anche di azioni che corrispondano all'interesse comune, ad una idea di compattezza e di unità. È proprio nei momenti più difficili che c'è bisogno degli sforzi e dell'azione coordinata dei Paesi con una forte tradizione europeista, più che di accordi bilaterali. È nei momenti più difficili che occorre dare nuovo slancio alla realtà politica, economica, sociale e culturale europea. L'Unione rappresenta ormai una realtà di diritto, cari colleghi, che nasce dalla volontà politica dei Governi degli Stati membri e dalla codecisione del Parlamento europeo, dove sono rappresentate le forze politiche nazionali: una realtà dalla quale sarebbe dannoso per tutti un ritorno indietro. Sarebbe un errore, un grave errore. Di fronte alla crisi globale, che ha messo in luce le contraddizioni e gli squilibri dell'idea ultraliberale, c'è bisogno che la politica torni in campo per restituire fiducia e speranza, indicare una prospettiva nuova di giustizia sociale e pari opportunità. Anche per questo ritengo che non giovi al Paese il gioco dello «scaricabarile»: l'Europa ci impone, l'Europa ci obbliga. L'Unione, nel quadro delle regole comuni, offre opportunità ai Governi degli Stati membri per la risoluzione coordinata dei singoli problemi. Merita, in questa sede, sottolineare che la nostra appartenenza all'Europa richiede un esercizio continuo di mediazione e integrazione tra interesse nazionale e interesse comune. Questo sospinge tutti gli attori politici verso una duplice responsabilità pubblica. Per quanto ci riguarda, abbiamo esercitato e vogliamo continuare ad esercitare questa responsabilità con impegno concreto, convinti come siamo che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia, soprattutto in questo momento, ha ancor più bisogno di Europa. Questo è stato il senso della nostra risoluzione alla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e degli emendamenti presentati alla legge comunitaria. Proposte concrete, per rendere il nostro rapporto con l'Unione più stringente, coerente e partecipato sia nella fase ascendente, che in quella discendente, anche per il rispetto dovuto al Parlamento, che è chiamato a svolgere un lavoro di adattamento all'ordinamento europeo non generico, ma puntuale e profondamente incardinato all'ordinamento nazionale. Abbiamo proposto a questo scopo di distinguere la legge comunitaria dalla Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: lo abbiamo fatto perché siamo convinti che in un sistema di *governance* multilivello come è quello europeo, abbiamo bisogno di entrambi i momenti, uno politico ed uno legislativo, adottando uno stile più inclusivo, cooperativo e interattivo. Infatti, favorire l'assestamento istituzionale ai nuovi compiti di costruzione, di recepimento e implementazione delle politiche europee, tanto nella fase ascendente che discendente, un imperativo democratico. In un'Unione di 27 Stati membri e quasi mezzo miliardo di abitanti, in un mondo sempre più complesso, non si può pensare che gli interessi nazionali siano difesi dai soli Governi. In questo quadro, le rappresentanze ai vari livelli devono poter concorrere non solo all'applicazione delle decisioni, ma anche alla elaborazione ed alla contrattazione comunitaria. Sempre di più il Parlamento è chiamato ad assolvere questo nuovo compito, in particolare attraverso le varie Commissioni che, con una seria e coerente revisione dei Regolamenti, devono essere messe in condizione di poter svolgere questa duplice funzione legislativa. La legge comunitaria 2008, come già i colleghi e le colleghe del mio Gruppo hanno avuto modo di dire, riveste per noi una particolare importanza per le direttive contenute che riguardano il completamento e il riposizionamento del mercato interno. Quello che voi non volete o fate finta di non voler capire è che queste direttive sono considerate, in Europa, le leve da azionare per reindirizzare la crescita, porre le premesse per uscire dalla crisi e raggiungere gli obiettivi dì Lisbona. E in questo modo sbeffeggiate il Paese: la direttiva servizi, per esempio, implica una grande liberalizzazione ed un complesso lavoro di attuazione a livello di Regioni, Comuni e, persino, di privati; richiede uno scambio coordinato e tecnologicamente avanzato con tutti gli Stati membri; e ci si vorrebbe far credere che tutto questo sia possibile con un'azione di recepimento solo formale, cioè a condizione che sia a costo zero! Siamo in presenza di una contraddizione che ha il marchio della resistenza passiva alle regole comuni. Una scelta questa che nel giro di poco tempo ha prodotto il ritorno alla frammentazione interna all'Esecutivo, la cancellazione di ogni idea di sussidiarietà, il disordinato processo di recepimento e la competizione fra Dicasteri. Per la direttiva sull'esercizio delle attività televisive, che ha lo scopo di adeguare la normativa allo sviluppo tecnologico e del mercato, avete fatto muro sugli emendamenti in difesa di interessi di parte. Tuttavia, apprezziamo l'ordine del giorno sulla tutela dei minori. In materia di cooperazione giuridica e di lotta alla criminalità organizzata, avete rifiutato anche emendamenti di buon senso, come la non violazione dei diritti fondamentali. Nel campo della parità uomo donna, abbiamo fatto proposte per recuperare al più presto la carenza tutta italiana nell'attuazione delle sette direttive sulla parità, oggetto in questa comunitaria, di refusione. Rispetto al quadro normativo europeo l'Italia, infatti, come è già stato ampiamente detto, è agli ultimissimi posti per parità retribuiva, per accesso al lavoro, per occupazione femminile, per rappresentanza e per tutele sociali. Ma svetta al primo posto per disoccupazione, per occupazione *part time* e per crollo delle nascite. Una situazione discriminatoria drammatica, nota a tutti, che ben si coniuga con la preoccupazione allarmata del commissario europeo Spidla che ha lanciato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione in cui chiede ai 27 Governi dell'Unione europea «di non continuare a sprecare il potenziale delle donne nell'economia, soprattutto in questo momento di crisi». crisi». Il dividendo sociale e democratico dell'investimento sulle donne è, ormai, evidente in tutta Europa. Ma non ancora nel nostro Paese. Con i nostri emendamenti ci siamo sforzati di contribuire a dare risposte a questa urgenza che chiama in causa un'etica redistributiva a voi sconosciuta perché troppi presi dal compiacere l'ansia ragionieristica del ministro Tremonti. Ma, in effetti, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza si configura come assai più grave perché lesivo del concetto di uguaglianza delle differenze. nel momento in cui il nostro Paese è chiamato a rispettare il principio di non discriminazione, su un punto ritenuto per anni il risarcimento delle donne per tutte le evidenti discriminazioni, ci si aspetterebbe uno sforzo congiunto per porre rimedio a tali discriminazioni, invece di spacciare obblighi giuridici per parità e per impegnarsi ad attuare un piano di azioni positive che ci avrebbe facilitato il prossimo recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea sul lavoro notturno. Ecco, questa è la discussione che va fatta e va fatta con mente serena, con spirito aperto e fuori da ogni logica di parte, nell'interesse delle donne e dei cittadini italiani tutti, che non devono avere una immagine distorta della nostra appartenenza all'Unione europea. L'Unione europea di oggi, infatti, è una tappa significativa di quel cammino intrapreso dai padri fondatori. L'Unione europea contemporanea è un insieme di diversità che nel passato ha creato tensioni e guerre, ma che oggi più di ieri rappresenta la vera forza per uscire dalla crisi dando energia all'economia mondiale, a robuste istituzioni democratiche ed a valori forti. signor Presidente, pur non condividendo le posizioni del Governo, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore dell'ordinamento europeo contenuto nella legge comunitaria e degli indirizzi programmatici contenuti nella Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

non fare, se possibile, capannelli in Aula. SANTINI vorrei annunciare subito, per non dimenticarmene alla fine nella foga del mio intervento, il voto favorevole e convinto del Popolo della Libertà sulla legge comunitaria.

consente ora, in sede di dichiarazione di voto, di alzare un po' lo sguardo su temi giuridici e politici di maggior contenuto, accanto a quelli tecnici. il rito di questa legge comunitaria consente ogni anno di allargare lo sguardo sulla problematica più vasta del processo di integrazione e coesione che l'Europa sta affrontando, quasi un esame periodico del suo stato di salute. Fra i molti temi che già sono stati trattati, ne vorrei richiamare uno di particolare attualità: la clausola di cedevolezza, che si riferisce al ruolo delle Regioni. Le Regioni sono al centro (al Senato lo sono già state e lo sono ora alla Camera dei deputati) del grande dibattito sul federalismo, ma esse sono protagoniste anche in Europa di un tentativo di ottenere un ruolo di di dialogo e di interlocuzione con le istituzioni europee. Bene, a tale proposito è utile ricordare che in Europa il dialogo interistituzionale avviene fra le istituzioni europee ed i Governi

quando, attraverso il comitato delle Regioni, hanno lasciato intendere che il loro intento non è soltanto quello di implementare le direttive e i regolamenti europei con la loro consulenza nei confronti della Commissione (questo è il compito del comitato in oggetto), ma che c'è un'ambizione un po' più vasta, quella di partecipare attivamente al processo legislativo, quasi alla pari con il ruolo del Parlamento europeo. Chiaramente tutto ciò non è accettabile, anche per ragioni di appesantimento di procedure ed allungamento del processo stesso. Va inoltre ricordata - la Corte di giustizia e la Corte costituzionale lo fanno quasi quotidianamente - la priorità dello Stato sulle Regioni ed il potere sostitutivo, sempre dello Stato, nei confronti delle Regioni; soprattutto laddove queste sono sono inadempienti scatta la clausola dell'infrazione comunitaria, che è a carico, per l'appunto, non delle Regioni ma dello Stato. Ferma restando la potenzialità della competenza di prima istanza delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di rispettiva competenza, è poi lo Stato che deve trattare con le istituzioni europee. Signor

di un'azione moralizzatrice nei confronti delle Regioni, invitandole a chiudere immediatamente tutte le sedi di rappresentanza a Bruxelles, che non servono più a nulla

oltre 600 Regioni: vi assicuro che i funzionari della Commissione europea sono disperati e quotidianamente assillati da richieste di interventi diretti di tutte le Regioni. Richiamino questi funzionari nelle rispettive sedi e, opportunamente istruiti, potremo copiare quello che fece la Spagna vent'anni fa, richiamando funzionari preparati a Bruxelles, in grado di dialogare dalle rispettive sedi di competenza. Chiudiamo queste istituzioni

di diventare soggetto di interlocuzione diretta anche sotto profili di politica estera e questo non è assolutamente accettabile. Questo vale naturalmente anche per molte altre attività, come quella della cooperazione allo sviluppo, in nome della quale molte Regioni e molte Province vanno in giro per il mondo a portare lodevolmente il frutto della solidarietà, ma anche a creare situazioni di profonda ambiguità.

allora recuperare un ruolo più credibile e una generale credibilità. L'Europa soffre, in fondo, di molti luoghi comuni: si dice che l'Europa è semi-impotente, che è tutta colpa dell'euro se c'è la crisi economica, e all'interno di questi luoghi comuni

a Durban 2, la Conferenza dell'ONU sul razzismo, tutti i Paesi europei hanno dichiarato di seguire l'esempio dell'Italia e del Ministro degli affari esteri italiano, che, coraggiosamente, per primo

Ricordo ancora, come credo tutti in quest'Aula, gli echi entusiastici della celebrazione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma:

momenti di titubanza vi sono sempre stati, lo diceva anche nel XIX secolo Alexis de Tocqueville, quando rammentava dopo avere ottenuta la liberazione, bisogna insegnare ai popoli a gestire la libertà: non dimentichiamo che in questa nuova Europa vi sono 12 Paesi di recente libertà. «L'uomo deve imparare a comprendere quanto sia stretto il legame del suo vantaggio personale con quello della collettività». Su questi presupposti, c'è un processo di coesione che sta avanzando ed è un processo che, anche tra l'indifferenza di molti Stati, fa grandi passi avanti. Questa legge sottolinea, accanto agli aspetti concreti e giuridici, i grandi passi in avanti

dello spazio di libera circolazione per le persone, per le merci e per i capitali. Sono aspetti non secondari che porteranno, speriamo, verso il completamento di quel processo, che appare ancora come un'utopia, delle comuni istituzioni politiche; è un progetto ancora ambizioso, ma sempre de Tocqueville ricordava: «L'uomo non può godere della libertà politica, se non a prezzo di molti sacrifici, e la ottiene sempre e solo con grandi sforzi». Dovremmo ricordarci di questi ammaestramenti anche in occasione di ricorrenze come questa, apparentemente tecnica e burocratica. Qualcuno, infine, signor

voi dite nell'Europa non c'è unità; neanche in Italia c'è unità, nemmeno in qualsiasi altra Nazione troverete l'unità psicologica, l'unità della convinzione religiosa. Ma, allora, qual è lo sforzo cui siamo chiamati oggi È il tentativo di creare una legge fondamentale di convivenza civile in cui tutti coloro che credono possono lavorare insieme per la ricostruzione del mondo. Questa legge l'avevamo creata, signor Presidente, si chiamava Costituzione europea. Ora è stata ridimensionata (e di molto) nel timido, pallido Trattato di Lisbona. Auguriamoci che almeno quello venga recepito da tutti gli Stati al più presto, magari prima delle elezioni europee. Infine, un' ultima considerazione. In Europa - lo sappiamo - si procede a piccoli passi,

i sogni piccoli - diceva Goethe - non hanno il potere di smuovere il cuore della gente. Potrà apparire perfino enfatico ed esagerato ricordare tutto questo in sede di discussione di una normale legge comunitaria che ha, ripeto, un carattere eminentemente tecnico e burocratico, ma tutto ciò aiuta a capire che l'Europa non è soltanto questo ma è anche, ancora una volta, l'occasione per rilanciare un sogno più ambizioso che coinvolge non solo i mercati, ma la crescita civile e democratica dei suoi cittadini. che sono presenti nelle tribune, in occasione della loro visita al Senato, gli studenti della 3a classe dell'Istituto tecnico commerciale in lingua tedesca di Bolzano «Heinrich Kunter», Kunter», accompagnati dal professor Oberhammer e dalla professoressa Geier. A tutti voi, come agli altri studenti che vengono a visitare il Senato, rivolgo i migliori auguri per la vostra attività di studio.

Passiamo ora all'esame della proposta di risoluzione n. 1, relativa alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, accolta dal Governo.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1078 e della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Ricordo che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun Gruppo ha a disposizione 20 minuti, comprensivi di illustrazione, interventi in discussione e dichiarazioni di voto. voto. Ha facoltà di parlare il senatore Tomassini per illustrare la mozione n. 93. Prego gli altri senatori di restare in silenzio o di uscire dall'Aula: questa è l'alternativa che si pone.

onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il tema dell'AIDS è molto noto a parole, ma molto poco conosciuto nei fatti e nei comportamenti. È pericolosissimo per la salute pubblica e diffusivo. È sicuramente contrastato in maniera opportuna dalle recenti scoperte e cure, ma sicuramente non è vinto.

I dati di arresto della malattia e della diminuzione del contagio non sono più così chiari come qualche anno fa. Proprio nel Lazio e nella Toscana emergono dati che segnalano una nuova ripresa dell'andamento epidemiologico.

Chi è sieropositivo tanto spesso non è consapevole di esserlo e questa mancanza di consapevolezza riduce i suoi diritti e anche quello spazio che sarebbe praticabile, pur nell'ambito del massimo di riservatezza.

identificando i gruppi di fragilità, predisponendo gli strumenti necessari e ben mettendo in luce quali devono essere gli standard di accesso

nei confronti di una malattia che sicuramente non è debellata e che rappresenta tuttora un grave pericolo diffusivo per la sanità pubblica. *(Applausi dai

L'anno scorso le conclusioni del Copenhagen Consensus, un *panel* composto da alcuni dei più importanti economisti a livello internazionale, hanno ammesso che la lotta all'AIDS è al primo posto nella lista delle priorità, giudicando l'eradicazione della malattia come l'intervento dai maggiori benefìci economici in termini assoluti. Negli ultimi anni si assiste ad un silenzio diffuso sull'infezione da HIV che contribuisce a sostenere l'idea, terribilmente sbagliata, che l'AIDS sia ormai prevalentemente un problema dei Paesi in via di sviluppo. È vero che in tali Paesi vive la maggior parte dei 40 milioni di persone malate di AIDS: in questi Paesi ogni minuto muoiono 7 persone e ogni giorno 17.000 contraggono il virus.

I più indifesi, di fronte a tale flagello, sono i bambini e gli adolescenti. Secondo i dati del Rapporto mondiale sull'AIDS 2008 delle Nazioni Unite, l'epidemia dell'AIDS ha provocato circa 2,1 milioni di vittime nel corso del del 2007, di cui 330.000 erano bambini, minori di quindici anni. Ogni minuto un bambino muore per cause collegate a questa malattia e quattro sono i nuovi contagi che avvengono tra gli adolescenti. Sono oltre 15 milioni i bambini nel mondo che hanno perduto uno o entrambi i genitori a causa di questa malattia. L'AIDS sta cambiando in modo radicale l'infanzia di milioni di bambini, privandoli dei loro diritti. Tale fardello, però, è in parte evitabile prevenendo la trasmissione dell'HIV da madre a figlio, provvedendo alle cure pediatriche, prevenendo il contagio tra gli adolescenti e i giovani, proteggendo ed aiutando i bambini colpiti da HIV. Il contrasto con il dramma dei Paesi più poveri è quello dell'Occidente, dove sono stati compiuti passi in avanti: assistiamo ad una diminuzione delle morti per AIDS, ma contestualmente anche ad un aumento del numero delle persone sieropositive. Questo dato è oggettivo e nei reparti ospedalieri sono sempre più le persone in cura. Cambiano anche in Europa le categorie colpite. Prima la malattia era particolarmente diffusa fra tossicodipendenti e omosessuali; oggi questa classificazione non è più valida: i sieropositivi sono soprattutto eterosessuali, e molto spesso donne. Aumenta anche l'età media delle persone colpite, perché si arriva fino a quarant'anni. Questo cambio del profilo rappresenta un chiaro segnale di una bassa percezione del rischio di questa malattia, soprattutto tra chi si infetta per via sessuale, e quindi ci dimostra come le campagne di sensibilizzazione e di prevenzione non siano state sufficientemente efficaci. Chi si infetta però oggi nel nostro Paese, in un Paese occidentale, ha una prospettiva di vita sicuramente maggiore (trent'anni) rispetto a quella

e la riduzione degli ostacoli alla sperimentazione, nonché di garantire un tempestivo trattamento e la comunicazione dei relativi benefici». benefici». Un'attenzione particolare, soprattutto in Italia, è da riservare agli immigrati. Dai dati forniti dal centro operativo AIDS dell'Istituto superiore di sanità emerge un aumento dei casi tra gli stranieri la cui proporzione è cresciuta dal 4,6 per cento del 1994 al 20,8 per cento del 2006. Il Registro nazionale dell'AIDS mette in evidenza un incremento della proporzione di malati di AIDS notificati tra i cittadini stranieri. Nel caso del contagio da HIV i migranti sembrano essere più esposti per la loro elevata mobilità e per il loro *status* legale che comporta scarsa informazione sull'accesso ai servizi sanitari di prevenzione. Gli stranieri non in regola che accedono alle cure sono sempre di meno e naturalmente il decreto sicurezza che avete approvato poco tempo fa, che costringe i medici a denunciare alle autorità giudiziarie gli immigrati clandestini, fa sì che gli immigrati malati di AIDS si Pertanto, il numero di questi malati aumenterà. È un atteggiamento, questo, che si scontra con la garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini, come vuole il nostro dettato costituzionale, approvata, che non favorisce di certo la prevenzione, anzi aumenta vertiginosamente i rischi. Non è possibile che persone malate debbano avere paura di essere curate. Vorrei a questo proposito ricordare al Governo che l'accesso alle cure è uno degli obiettivi che l'Italia, insieme ai Paesi del G8, si è impegnata a garantire entro il 2010 per contrastare la diffusione dell'HIV, della malaria e della tubercolosi. L'impegno che chiediamo al Governo è un impegno chiaro che non può non essere condiviso, cioè quello di realizzare un piano di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dell'AIDS, approntando misure specifiche, in particolare, per la tutela dei minori sieropositivi; stanziare risorse idonee per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili, proprio nel rispetto della risoluzione del Parlamento europeo; realizzare un sistema di diagnosi precoce dell'infezione da HIV, anche nei confronti dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla condizione di regolarità o meno del loro soggiorno; garantire un costante monitoraggio in ordine alla diffusione del virus dell'HIV nell'ambito della popolazione presente sul territorio nazionale; realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione di questa malattia, favorendo, tra l'altro, l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole; adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti malati di

che affrontano la complessità delle problematiche legate alla lotta all'AIDS, c'è un comune denominatore: la piena consapevolezza da parte di tutti della gravità e drammaticità, sul piano umano, sanitario e sociale, che il fenomeno dell'AIDS ricopre nel nostro Paese e in ogni angolo del mondo. Questa consapevolezza non ci viene solo dalla conoscenza dei numeri, in valori assoluti, che delineano l'entità della diffusione di questa piaga: solo in Italia - e sono dati del Ministero della salute - dall'inizio dell'epidemia al dicembre 2007, si sono registrati 58.000 casi di AIDS e, tra questi, i decessi sono stati 35.000. Ma la consapevolezza proviene anche dall'impatto che le dimensioni globali dell'epidemia stanno producendo sull'infanzia e sull'adolescenza, con stime in costante evoluzione: nel 2007, se guardiamo alle stime globali sulla pandemia, 2 milioni di persone sono morte per cause correlate all'AIDS e, di queste, 290.000 erano bambini sotto i quindici Se a questo poi aggiungiamo i dati dell'UNICEF e dell'Agenzia ONU, appare sconcertante l'allarme che soltanto il 10 per cento dei bambini sieropositivi riceve cure adeguate, e che, di questi, circa 4 milioni necessitano del cotrimoxazolo, un semplice antibiotico facilmente reperibile, che costa solo pochi centesimi di euro al giorno per bambino, antibiotico che può prevenire le infezioni a volte letali e ritardare i sintomi dell'AIDS. Questo ci dà la percezione della complessità del tema che oggi stiamo trattando. Sono significative al riguardo non solo le due risoluzioni del Parlamento europeo, richiamate nelle nostre mozioni, quella dell'aprile 2007 e quella del novembre 2008, nella quale si sottolinea l'importanza di introdurre misure efficaci di salute pubblica, volte a facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da virus HIV; ancor più significativa, anche nel suo titolo, è la risoluzione che il Parlamento europeo approvò in data anteriore, nel luglio 2006, alla quale intese dare un titolo particolarmente esplicativo con le parole «Tempo di agire». È tempo di agire perché non ci sono più categorie a rischio, ma popolazioni vulnerabili. È tempo di agire perché i risultati rimangono ancora insufficienti, sia sotto il profilo della prevenzione, che della disponibilità delle terapie, a fronte dell'impegno assunto dai vari Stati di garantire una copertura del 100 per cento, entro il 2010, dei farmaci salvavita, obiettivo che abbiamo chiamato dell'accesso universale, che oggi raggiunge solo il 30 per cento di coloro che ne hanno bisogno. Che si debba fare qualcosa di serio, anche nel nostro Paese, con un'attenta programmazione e un capillare monitoraggio, ce lo dicono due dati apparentemente contrastanti, ma che danno l'esatta comprensione delle responsabilità che ci attendono. Il primo dato è la diminuzione di mortalità: a partire dal 1997 si inizia a registrare un progressivo decremento; questo significa che è possibile ottenere una diminuzione di mortalità che essa è anche e soprattutto conseguenza diretta del progressivo inserimento nella pratica medica delle nuove terapie antiretrovirali. Il secondo dato, che ci fa apprezzare il valore della diagnosi precoce, è che oltre il 60 per cento dei casi di AIDS registrati in Italia si verifica in persone che non hanno fatto terapie prima della diagnosi e ciò è dovuto al fatto che sempre più persone (oltre il 50 per cento) scoprono di essere sieropositive a ridosso della malattia conclamata. In Italia almeno 130.000 persone sono sieropositive, mentre i casi diagnosticati sono soltanto 65.000. In parole semplici, l'Istituto superiore di sanità stima che il 50 per cento dei sieropositivi presenti in Italia siano soggetti non identificati. Ecco perché il problema non è più rimandabile. Ecco perché vi è l'allarme che, nonostante l'evidenza scientifica del buon funzionamento di alcuni interventi di prevenzione, molti Governi - tra cui anche il nostro - ancora non li applicano. Ed ecco perché, nella nostra mozione, noi proponiamo un modello di prevenzione combinata, sia attraverso l'adozione di un piano nazionale volto a promuovere l'accesso all'educazione e all'informazione, sia attraverso l'avvio di programmi concreti rivolti in modo particolare alle fasce giovanili. La prevenzione di cui abbiamo bisogno oggi, alla luce delle conoscenze attuali, è un intervento ampio, basato su una combinazione integrata di approcci e strumenti che vanno dalle tecniche biomediche agli interventi comportamentali. Nella nostra mozione abbiamo voluto inoltre sottolineare, in maniera responsabile, con un forte richiamo al Parlamento e al Governo, le gravissime conseguenze che nella lotta alla malattia del secolo si potrebbe avere dall'allontanare ulteriormente i cittadini stranieri irregolari dal contatto con il servizio pubblico ospedaliero. Per questo impegniamo il Governo ad attuare un piano di prevenzione per facilitare l'accesso al *test* di diagnosi precoce anche nei confronti di cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno dei loro soggiorni. Noi impegniamo il Governo a rivedere il disegno di legge sulla sicurezza, in discussione alla Camera dei deputati, che prevede la cancellazione del divieto di segnalazione per gli immigrati senza permesso di soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie per curarsi, perché la sola possibilità e non l'obbligo di denuncia può produrre effetti devastanti sia per gli immigrati che per tutti i cittadini italiani. Oggi, alle ore 18, in venti città italiane sono state organizzate manifestazioni da parte di associazioni mediche e di operatori sanitari, contro la facoltà di denuncia alle autorità per i pazienti immigrati irregolari che si rivolgono a una struttura sanitaria. È una norma contraria all'etica È una norma contraria all'etica e alla deontologia medica, contraria al vincolo del segreto professionale e al dettato costituzionale che tutela la salute individuale e collettiva; è una norma che, alla luce delle problematiche che sono oggetto della nostra mozione, va va contro ogni criterio di buonsenso perché gli stranieri non in regola, per timore di essere identificati ed espulsi, non si cureranno o lo faranno in strutture non riconosciute e ci si esporrà sempre più al rischio di diffusione di malattie. In ultimo, nella nostra mozione impegniamo il Governo a stanziare adeguate risorse per favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi trattamenti delle patologie sessualmente trasmissibili e dell'AIDS; e, soprattutto, a mantenere gli impegni assunti a livello internazionale, volti a realizzare l'accesso universale, aumentando l'impegno finanziario da destinare al fondo globale per la lotta all'AIDS. Non vanno ripetuti gli errori fatti a metà degli anni quando HIV e AIDS sono usciti dall'agenda politica di molti Governi e il virus ha potuto diffondersi indisturbato, causando morti e malattie.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Bosone per avermi dato parte del suo tempo per questo intervento. Io sono, insieme alla senatrice Poretti, uno dei cofirmatari della mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico. Ho ritenuto di dover arricchire parte di ciò che viene presentato in quel documento perché, secondo noi (non abbiamo avuto il tempo di tradurre questi nostri suggerimenti in paragrafi),

dagli studi sul virus dell'HIV e sull'AIDS, la sua conclamazione, e si è passati dal parlare di categorie di persone a veri e propri comportamenti.

sociosanitarie che passano sotto il nome di riduzione del danno. Noi siamo a favore di questo documento, ma vorremmo che il Governo, in maniera chiara, dicesse cosa pensa relativamente alle siringhe sterili alla possibilità di somministrazione controllata di sostanze stupefacenti incluse nelle tre Convenzioni delle Nazioni Unite, perché anche queste misure

mozioni sono estremamente importanti proprio per mantenere alta la vigilanza ma anche per suggerire nuovi interventi, che si impongono vista la diversa epidemiologia attuale della malattia. una malattia ormai endemica anche nella nostra Nazione, come in Nord America, e non più epidemica come in altre zone quali l'Africa. alcune osservazioni, che traggo soprattutto dalla realtà sanitaria della mia Regione, la Val d'Aosta. È chiaro che i farmaci e la terapia antiretrovirale hanno permesso una sopravvivenza maggiore di questi malati e un maggior controllo della malattia; aumentando però il numero dei malati, che

signor Ministro, un'alta vigilanza su questo problema proprio perché la malattia è trasmissibile e i malati sono più numerosi. Si impongono anche nuove strategie, come la diffusione del test prevista

Presidente, svolgo alcune brevi considerazioni su queste mozioni. mozioni. Una prima considerazione che va sicuramente fatta è che, dopo l'iniziale allarme, al momento di comparsa della malattia, al momento dei primi contagi e al momento nel quale si è visto che l'infezione galoppava e quindi vi è stato un

il momento che sembrava culminante e nel quale anche l'informazione seguiva molto l'argomento, si è persa, sostanzialmente, tutta questa attenzione. Quindi, per queste mozioni che riportano l'attenzione del Parlamento, e del nostro Paese in particolare, su questo argomento.

che, quantomeno, tengono la malattia in quiescenza e ne diminuiscono il danno. Io credo, però, che in tutte le mozioni non sia stato messo sufficientemente in risalto il fatto

veramente carenti, è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Noi dobbiamo sicuramente insegnare ai nostri ragazzi che non devono buttarsi via e che quindi un rapporto sessuale non dovrebbe essere occasionale, fatto tanto per fare qualcosa, ma dovrebbe seguire ad una spinta ideale e affettiva.

insegnare alle persone che devono volersi bene, devono avere rispetto per se stesse e dunque devono difendere

hanno sottolineato il fatto che nel decreto sicurezza è stato approvato un emendamento

un discorso diverso e un po' più complicato, per quanto riguarda la tubercolosi voglio ricordare che le motivazioni per cui è necessaria la segnalazione sono proprio quelle di tutela della salute della società. A me hanno insegnato, quando studiavo

scusate, ma come potete pensare di portare avanti trattamenti lunghi come quelli che servono ad esempio per la tubercolosi - il cui trattamento deve durare sei mesi

È esattamente tutto il contrario di quello che affermano in questi giorni molti medici! A questo punto questo punto voi potreste chiedermi se vale di più la tutela dell'individuo o la tutela della società in cui vive l'individuo dal punto di vista sanitario. Secondo me, va tutelato l'individuo, perché va curato, ma se l'individuo è fonte di trasmissibilità e di infezione va tutelata anche la società e quindi

Ritorno all'AIDS: credo ci sia veramente bisogno di un ritorno all'attenzione su questo tema e di un ritorno alle cure, soprattutto per i minori.

e credo che ci debba essere anche qui da noi un grande impegno, anche, come ho detto, a riportare l'attenzione delle persone su questo che è e rimane un pericolo grandissimo. *(Applausi

Presidente, colleghi, sul problema dell'HIV e dell'AIDS vi è stato in questi anni un calo di attenzione, non solo e non già della comunità scientifica e medica, ma soprattutto della comunità politica e sociale,

prevenire anche tra di loro, negli ambiti dei centri di prima accoglienza in accordo, a mio avviso, con le associazioni umanitarie che si occupano di immigrazione e di accoglienza di immigrati. court*, regolari e irregolari, perché dentro il fenomeno dell'immigrazione risiede il vero problema dell'attuale aumento dei sieropositivi e della diffusione dell'infezione, soprattutto tra questa popolazione molto debole e fragile. È chiaro che l'immigrato va inserito e accolto nel sistema sanitario nazionale. Spero e mi auguro quindi che questa mozione sia prodromica al fatto che alla Camera il centrodestra

responsabile e una assunzione di responsabilità da parte dei giovani, portandoli a conoscenza dei rischi veri insiti in un rapporto occasionale. Spero che queste mozioni possano essere viste in modo complementare, perché ci aiutano a riportare il problema AIDS al centro della nostra attenzione.

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'HIV/AIDS è un grave problema di sanità pubblica e i dati aggiornati del rapporto 2008 sull'epidemia di AIDS, presentati dal programma congiunto delle Nazioni Unite e dell'OMS, ne sono la prova: si stima che nel 2007 siano 33 milioni le persone affette da HIV, 2,7 milioni quelle che hanno appena contratto il *virus* e 2 milioni i malati deceduti per AIDS. L'infezione da HIV/AIDS è molto diffusa in Europa e i dati della relazione di fine anno per il 2006 indicano che nel periodo 1999-2006 le persone che hanno contratto il *virus* dell'HIV sono state più di 269.000 all'interno dell'Unione europea

Il numero di nuovi contagi HIV continua a crescere ad un tasso preoccupante nell'Unione europea e nei Paesi vicini e in alcuni Paesi il numero di persone che si stima siano contagiate dall'HIV è di quasi tre volte superiore alle cifre ufficiali; un'elevata percentuale di infezioni da HIV rimane non diagnosticata e molte persone non sanno di essere infette e con ogni probabilità lo scopriranno soltanto una volta colpite da malattie connesse con l'HIV/AIDS; l'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di altre malattie a trasmissione sessuale: mi rifaccio all'importanza di insegnare ai nostri ragazzi di avere rapporti protetti, senza vergognarsi di chiederlo e di pretenderlo. L'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di queste malattie a trasmissione sessuale. L'epidemia tra i consumatori di droghe iniettive è una delle cause della rapida diffusione dell'infezione da HIV in numerosi Paesi dell'Europa orientale. in Italia non è certamente più rosea: i dati degli ultimi sei mesi di monitoraggio dell'infezione effettuato dal Centro Operativo AIDS dell'Istituto superiore di sanità (COA) e pubblicati a dicembre 2008 illustrano un quadro in cui l'infezione rimane costante e non diminuiscono certamente i casi. Le stime elaborate per il 2008 presentano oltre 5.600 nuovi casi di AIDS in Italia e circa 130.000 nuove infezioni da HIV. Dall'inizio dell'epidemia le infezioni in Italia sono state tra 140.000 ed i 180.000, i casi di AIDS si attestano attorno a più di 60.000, con 39.000 morti circa. Negli ultimi tre anni si sono registrati sempre in Italia circa 4.000 nuovi casi di contagio l'anno, con un'incidenza maggiore tra gli eterosessuali. C'è, purtroppo, in generale - come è giù stato sottolineato ma mai abbastanza - una bassa percezione del rischio, per cui sono sempre più numerosi coloro che scoprono di essere sieropositivi nel momento in cui hanno la diagnosi di AIDS:

accadeva in passato, ma persone che hanno contratto il *virus* HIV per via sessuale (per contatti eterosessuali nel 44,4 per cento dei casi e omo-bisessuali in più stranieri (oltre il 20 per cento dei casi). E se un tempo il *virus* HIV colpiva soprattutto i giovani tra 20 e 30 anni, oggi la malattia colpisce in media persone tra 30 e 40 anni. significa che quasi il 60 per cento dei casi di AIDS scopre di essere sieropositivo poco prima o al momento della malattia conclamata, e questo suggerisce che la percezione del rischio è ulteriormente diminuita. più di 60.000 i casi di AIDS dall'inizio dell'epidemia, di cui oltre 20.000 viventi. C'è una lieve tendenza alla ulteriore flessione dell'incidenza di malattia conclamata, grazie alle terapie. dei casi di AIDS non ha fatto terapia prima della diagnosi. A fronte di questi recenti dati, è necessario sottolineare l'importanza del pericolo dell'HIV e non bisogna dimenticare quanto sia un serio problema per la salute pubblica; dobbiamo continuare a migliorare la conoscenza, la consapevolezza e soprattutto l'informazione sull'HIV-AIDS, specialmente tra i giovani e i gruppi a rischio. poiché la diagnosi tardiva porta a cura tardiva e quindi ad una minore qualità della vita per le persone che vivono con l'HIV-AIDS, è importante sottolineare la diagnosi precoce attraverso il *testing*. Le persone devono essere rassicurate sul fatto che conoscere il loro stato di salute li aiuterà, alla lunga, nella cura, e devono comprendere l'importanza per la loro vita dell'accesso precoce alla cura. Ricordando che l'HIV-AIDS è una malattia trasmissibile e che vi è quindi un rischio di contagio provocato dalle persone infette non diagnosticate, si pensa necessario garantire l'accesso al test. Inoltre, si ritiene opportuna la necessità di garantire un accurato monitoraggio ed una stretta sorveglianza da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tra cui stime più precise (per quantità, caratteristiche eccetera) della popolazione non diagnosticata, pur sempre nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Si dovrebbero anche impegnare sostanziali risorse politiche, umane e finanziarie per sostenere l'attuazione di tale strategia.

elaborare raccomandazioni sull'attuazione di sperimentazioni ed orientamenti in materia di trattamento fondati su dati comprovati in ciascuno Stato membro, nonché garantire che, in futuro, il monitoraggio dei progressi nella lotta contro l'HIV-AIDS in Europa e nei Paesi vicini comprenda indicatori che riguardano e misurano direttamente le questioni legate ai diritti umani. È infine necessario ricordare che vi è assoluta necessità di cooperazione transfrontaliera per affrontare l'epidemia. Con queste premesse, lo scorso novembre ha visto una particolare attenzione alla politica ed alla strategia messe in atto dalle istituzioni europee per la lotta all'AIDS. Il punto focale di questa attività è stata la «risoluzione del Parlamento europeo sull'HIV/AIDS: diagnosi e trattamento precoce», del 20 novembre dell'anno scorso. Attraverso questa risoluzione, il Parlamento europeo chiede una strategia volta a promuovere diagnosi precoce e tempestivo trattamento dell'HIV, garantendo l'accesso ai test ed un accurato monitoraggio; esso sollecita inoltre un strategia di riduzione dell'infezione e campagne di informazione ed educazione sulla prevenzione. Auspica poi raccomandazioni sull'attuazione delle sperimentazioni e chiede ai Governi di dichiarare illegale le discriminazioni contro persone affette dal virus, come le restrizioni alla libera circolazione.

i molteplici aspetti che caratterizzano il problema della persistenza e diffusione del virus HIV, in data 21 gennaio 2009, ho ricostituito la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, al fine di definire una strategia aggiornata, con valenza nazionale ed europea, nell'ambito della ricerca e della prevenzione, unitamente alla verifica dell'evoluzione del trattamento terapeutico. In tale sede, pertanto, verranno attentamente valutate tutte le iniziative attinenti all'AIDS, la cui necessità e urgenza le mozioni hanno evidenziato, come la facilità all'accesso al *test* diagnostico, linee-guida, lotta alla discriminazione, sviluppo della ricerca, informazione ai cittadini, con particolare riguardo al mondo dei giovani, procedure standard per l'accettazione e ricovero ospedaliero e per l'accoglienza di altri soggetti in stato di disagio sociale.

Grazie